Signor Presidente, l'articolo 165 del nostro Regolamento prescrive che sia il Presidente della 5a Commissione a esaminare il progetto di bilancio e il conto consuntivo, insieme con i Presidenti delle altre Commissioni, e a riferirne all'Assemblea. Progetto di bilancio e conto consuntivo che, com'è noto, sono predisposti dal Collegio dei senatori Questori e approvati dal Consiglio di Presidenza. Ieri sera c'è stata la riunione dei Presidenti delle Commissioni con i senatori Questori, il progetto di bilancio del 2016 e il conto consuntivo del 2015 sono stati esaminati

Nel provare a riferire sommariamente le considerazioni che insieme abbiamo elaborato, vorrei partire da

e che può essere un po' definito l'atto fondativo di un nuovo corso nella gestione delle risorse che la finanza pubblica mette a disposizione del Senato come della Camera dei deputati. Questo nuovo corso è stato, a mio modo di vedere, brillantemente incarnato dal Collegio dei Questori e dalle manovre di bilancio realizzate in questi anni e in questa legislatura. Mi riferisco all'ordine del giorno G100 del 3 agosto 2011, quindi nella XVI legislatura; nell'estate terribile della più grave crisi finanziaria, della finanza pubblica in modo particolare, che il nostro Paese ricordi dal dopoguerra in avanti, la famosa estate dello *spread* (pochi mesi dopo sarebbe caduto il Governo Berlusconi sostituito dal Governo Monti). Eravamo quindi in una situazione di grande tensione politica, sociale ed economica.

Finocchiaro, Bricolo ed altri, individuava un preciso programma di ristrutturazione e di riorganizzazione della spesa a disposizione del Senato, partendo proprio dalla situazione del Paese, con un richiamo forte al senso di responsabilità e di coerenza dei parlamentari e dei Gruppi politici. individuava un programma fatto di tagli alle spese ed introduceva un contributo di perequazione ai vitalizi, tagli alle retribuzioni più elevate, il blocco dell'adeguamento delle indennità e dei vitalizi dei senatori, una razionalizzazione del patrimonio immobiliare, interventi volti a stabilizzare nel tempo e a rafforzare il *trend* di riduzione della spesa complessiva. In particolare, esso individuava tre grandi questioni strutturali sulle quali intervenire: in primo luogo, distinguere e mettere in evidenza la spesa previdenziale rispetto al resto della spesa di funzionamento; una revisione della spesa, introducendo il concetto di bilancio a base zero, cioè la rimotivazione di tutto il sistema delle spese superando, con un po' di ottimismo della volontà (poi sappiamo che le cose sono sempre più difficili da farsi di quanto si vorrebbe realizzare), il bilancio sulla base della spesa storica; luogo, la progressiva integrazione di funzioni e strutture amministrative dei due rami del Parlamento. il progetto di bilancio 2016 e il rendiconto 2015 che ci viene presentato dai senatori Questori, che poi lo illustreranno in dettaglio, e che è stato approvato dal Consiglio di Presidenza, presenti risultati assolutamente rilevanti ed importanti. In particolare, vorrei evidenziare un dato fondamentale che è quello della spesa a consuntivo, che scende dai 520 milioni del 2012 ai 495 milioni del 2015. È raro trovare una amministrazione che riduca la spesa in termini nominali e a consuntivo. Spesso si chiamano riduzioni di spesa gli obiettivi di riduzione dell'aumento tendenziale. In questo caso, stiamo parlando di riduzione della spesa nominale,

Il progetto di bilancio mette in evidenza anche i vincoli con i quali i senatori questori devono operare, che sono

ovviamente con una certa fatica. Ebbene, penso che si possa dire che la tendenza verso la quale andiamo, che è confermata

Se andiamo a vedere le quattro voci fondamentali, più importanti e anche politicamente più sensibili, diciamo così, delle spese di funzionamento, vediamo che c'è un leggero

c'è un forte calo nella spesa per il personale, il che vuol dire che aumenta la produttività del lavoro in Senato e aumenta anche l'impegno dei nostri collaboratori e del personale a tutti i livelli (si passa dai 123 milioni del 2013 ai ai 102 milioni del 2015) e c'è invece una dinamica diversa della spesa previdenziale. Abbiamo un calo, sia pure modesto ma significativo, spesa per gli ex senatori (si passa dagli 80 milioni del 2013 ai 78 del 2015) è c'è invece un aumento significativo della previdenza per il personale che è in qualche modo anche l'altra faccia della riduzione della spesa corrente per il personale in servizio. È chiaro che incentivare il personale ad uscire comporta poi un aumento della spesa previdenziale. Questo è un elemento strutturale di preoccupazione sul futuro della struttura del nostro bilancio, perché abbiamo un calo complessivo della spesa di funzionamento che passa dai 309 milioni del 2013, ai 293 del 2014 e ai 272 del 2015, riducendosi sensibilmente, e un efficientamento complessivo della macchina, e parallelamente abbiamo una crescita della spesa di natura previdenziale, che va da 203, a 207, a 223 milioni nel 2015, con un'incidenza che passa dal 40 per cento del 2013 al 45 per cento del 2015. Questo *trend* porterà, nel giro di qualche anno, ad un pareggio tra le due voci o addirittura ad un sorpasso da parte della spesa previdenziale. Osservando Osservando il bilancio - ne ho parlato ieri anche con i colleghi Presidenti - non posso che consegnare all'Assemblea e naturalmente, innanzi tutto, al Presidente, la valutazione circa l'opportunità e la praticabilità di un intervento di natura strutturale su questo aspetto, promosso appunto dalle Presidenze di Senato e Camera di concerto con gli altri organi costituzionali e con il Governo, volto alla creazione di un ente di previdenza cui conferire una parte del patrimonio: le passività, cioè i trattamenti previdenziali, e le attività, cioè i contributi e i trasferimenti da parte dello Stato. Questo per liberare in prospettiva il bilancio del Senato e della Camera, ossia il bilancio del Parlamento, da una voce così pesante e significativa. Concludo con un'ultima notazione: credo che si sia avviato in questi anni in maniera molto positiva un lavoro di integrazione delle strutture tra Camera e Senato.

di affrontare non più soltanto dal punto di vista della politica del bilancio, ma con interventi di tipo strutturale il tema dell'uso ottimale delle risorse che il Paese mette a disposizione di Camera e Senato.

Signor Presidente, cari colleghi, portiamo all'attenzione dell'Assemblea il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e il rendiconto per l'esercizio 2015. Come negli anni passati, il Senato non si è minimamente sottratto, in un momento che rimane di grande difficoltà economica per tanti italiani, nonostante i primi timidi segnali di ripresa, all'impegno che accomuna tutto il Paese finalizzato al miglioramento dei conti pubblici. Entriamo adesso un po' più nel dettaglio delle voci dei due documenti che andiamo ad analizzare e che illustrerò brevemente. Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Tonini della sua illustrazione

Credo che questo sia un risultato veramente importante per quello che riguarda la spesa del nostro Senato e, addirittura, vorrei dire che i primi sei mesi del 2016 ci lasciano

di Palazzo Madama in termini di cassa si riduce quindi di 5,8 milioni di euro e si tratta di un livello di spesa che equivale a quello di dieci anni fa. Nel complesso, la spesa effettiva effettiva del Senato si è ridotta quasi del 5 per cento (precisamente 4,83) dall'inizio di questa legislatura. La dotazione è la voce principale delle entrate del Senato, che si attesta a euro 505.360.500. Il Senato quest'anno chiude in attivo, con un avanzo di esercizio di 44 milioni di euro.

Questa fetta del *budget* di Palazzo Madama, come vedete, è in netta diminuzione, mentre, dall'altra parte, la spesa previdenziale si attesta al 45,1 Nel passare in rassegna i principali eventi gestionali dell'esercizio 2015, a cui si riferisce il rendiconto, segnalo gli 11 milioni di euro da restituire al bilancio dello Stato come risultato dei risparmi di spesa ottenuti nel 2014, e le economie realizzate, pari a 4,4 milioni di euro, per effetto, appunto, delle decisioni del Consiglio di Presidenza in materia di retribuzioni. Sempre dando un rapido sguardo alle altre voci di spesa, vi segnalo che il trattamento del personale addetto alle segreterie particolari istituzionali ha registrato, nel biennio 2014-2015,

Sulla stessa scia è anche il capitolo degli ex senatori cessati dal mandato, che subisce un'ulteriore diminuzione di circa il tre per cento. Per quanto concerne l'assistenza sanitaria, il bilancio anche in questo caso è positivo: nel 2015 si registra un avanzo

Sul fronte del personale dipendente, si conferma un *trend* positivo, con una riduzione degli stipendi pari al 14,13 per cento; si passa da 123 milioni di euro a 102 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Di riflesso, diminuiscono chiaramente gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione: -2,5 milioni di euro rispetto al 2014, quasi -6 milioni rispetto al 2013. riguarda, invece, le spese relative ai servizi, le forniture e il funzionamento dell'istituzione, il Senato registra nel 2015 un'ulteriore diminuzione di 3,8 milioni, pari all'8,66 per cento rispetto al 2014, e una diminuzione di 8,8 milioni,

Le uscite ammonteranno a 544 milioni di euro, al netto dei risparmi da riversare allo Stato. Ancora una volta, il Senato riduce la propria spesa per il sesto anno il che significa che, da un punto di vista finanziario, il Senato si alleggerisce grazie ad una serie di azioni messe in campo che mirano, appunto, al contenimento della spesa.

da un lato, c'è la minore dotazione, che è un dato strutturale, e cioè le minori risorse richieste allo Stato; dall'altro, i risparmi aggiuntivi che, grazie ad un migliore impiego delle risorse e a un contenimento delle spese, siamo riusciti a conseguire. Dai dati strutturali si evince una minore dotazione dallo Stato, che si riduce ogni anno di 21,6 milioni di euro: quindi dal 2013 ad oggi registriamo un segno negativo di 86,4 milioni di euro che Palazzo Madama ha chiesto in meno allo Stato italiano. Dall'altro lato, in parallelo, ci sono due risparmi aggiuntivi e ciò significa che in questi anni, dal 2013 ad oggi, oltre agli 86,4 milioni di euro di minore dotazione, il Senato, grazie agli sforzi messi in campo, restituisce allo Stato ulteriori 65,5 milioni di euro. Pertanto, in un contesto complessivo, il peso

per effetto delle scelte del Consiglio di Presidenza in materia di retribuzioni, sono conseguiti risparmi pari a 6,2 milioni di euro per il 2016 che produrranno complessivamente un risparmio pari a 36,7 milioni di euro sempre per quanto riguarda i dipendenti. A questi primi due dati si aggiunge un dato tendenziale che riguarda invece la dinamica delle retribuzioni, che anche nel caso specifico cala, rispetto al 2011, di circa il 30

stiamo cercando in tutti i modi di procedere congiuntamente alla Camera per arrivare a una centrale unica di committenza, come prevedono le nuove normative. Credo che questi siano aspetti fondamentali per far sì che il Parlamento, nella sua complessità,

altro aspetto è la lotta allo spreco alimentare.

assicurare la qualità della spesa vuol dire anche lottare contro lo spreco alimentare nei settori della distribuzione e della ristorazione. Passo al settore della stampa e della prestampa digitale e della digitalizzazione. Anche su questo fronte il Senato ha fatto grandi passi

- del personale intervenuta. Sul fronte delle infrastrutture informatiche, Palazzo Madama dallo scorso anno ha puntato sull'innovazione. Il Senato è dotato delle tecnologie di virtualizzazione delle postazioni di lavoro e diventa così un modello per grazie a tutti proprio per questo, in relazione ai risparmi che derivano dai servizi di stampa digitale e dalle nuove infrastrutture informatiche,

penultimo Consiglio di Presidenza, ha voluto con forza ribadire che il processo di integrazione tra i due rami del Parlamento è partito all'inizio della nostra legislatura, al di là di qualsiasi modifica costituzionale. È partito con la prima delibera del 2013.

stiamo proseguendo con forza con questo nostro impegno. Vorrei oggi dire ai colleghi e agli amici dell'altro ramo del Parlamento dobbiamo fare presto perché raggiungere questo obiettivo significa dare anche una risposta concreta a tante domande che i cittadini si pongono rispetto alle strutture, all'amministrazione e all'organizzazione interna.

di armonizzazione - uso un termine impiegato in questi mesi - delle regole di contabilità e di redazione di un bilancio integrato che dia evidenza contabile ai risparmi conseguiti dallo svolgimento delle attività in comune. Ho letto questa frase per non

grazie a tutti

5 Stelle riguardano la cessazione, la decurtazione, la non cumulabilità, nonché l'adeguamento al sistema contributivo, al fine di abolire una vergogna nazionale.

ricchi premi dati alla classe politica che ha ucciso il nostro Paese. Dieci milioni di italiani sono sotto la soglia di povertà; trecentottanta imprese al giorno; un pensionato su tre prende meno di 1.000 euro al mese; e qui dentro si spendono 83 83 milioni di euro all'anno per ingrassare chi è già abbondantemente grasso. I politici italiani dovrebbero riconsegnare ai cittadini i soldi percepiti dallo Stato, per i disastri commessi; ma viceversa gli stessi italiani, da loro annientati, pagano a questi signori vitalizi pazzeschi, al di fuori di ogni logica e di ogni sostenibilità finanziaria. 1.899.925 pensionati percepiscono meno di 499 euro al mese; 4.731.779 pensionati percepiscono tra 500 e 999 euro al mese. E qui dentro vitalizi, prebende e rendite a sbafo. Per aumentare le pensioni minime i soldi non ci sono mai; per i vitalizi ci sono sempre. Le persone normali vanno in pensione sempre più tardi, perché i soldi non ci sono mai; per i vitalizi ci sono sempre. La giustizia è al collasso, perché non ci sono i soldi; per i vitalizi ci sono. La sanità ci distrugge, perché i soldi non ci sono; per i vitalizi ci sono. Per i cittadini i soldi non ci sono mai; per loro si trovano sempre, per i politici il piatto è sempre ricco. È giustizia questa secondo voi? È giustizia? I cittadini sono tutti uguali, dice la Costituzione, ma alcuni hanno il vitalizio e altri muoiono di fame. I risparmi della riforma costituzionale Verdini-Boschi possono essere raggiunti senza stravolgere la Costituzione repubblicana, in un battibaleno. Sapete come? Votando anche uno solo degli ordini del giorno del Movimento 5 Stelle. Con un solo voto oggi possiamo risparmiare di più di quello che risparmiamo con la riforma massonica che volete approvare. Con un solo voto, 83 milioni di euro l'anno potrebbero uscire da questi palazzi dorati ed entrare nelle tasche dei cittadini più poveri di questo Paese. L'abolizione dei vitalizi parlamentari non è solo parte integrante della missione che il Movimento 5 Stelle ha, ma è ciò che tutti gli italiani, ad eccezione di chi percepisce il vitalizio, chiedono a gran voce; e noi qui siamo quella voce. Oltre alla soppressione integrale dei vitalizi, pretendiamo quanto meno una loro riduzione in relazione alla situazione del Paese e soprattutto in relazione alla legislazione vigente. Poiché - ne sono certo - vi trincererete dietro l'incostituzionalità della soppressione integrale dei vitalizi, vorrei informare l'Aula che la Corte costituzionale ha recentemente ritenuto compatibile con il dettato costituzionale il cosiddetto contributo di solidarietà sulle pensioni di importo più elevato, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato dalla crisi contingente e grave del sistema. Dunque, se proprio non riuscite ad abolire i vitalizi, almeno un minimo cenno di dignità datelo ai cittadini. Ma sono certo che non voterete un bel nulla, come avete sempre fatto in questi anni. Quindi, onorevoli colleghi e cari senatori, vi ricordo che il vitalizio è atrocemente indegno sul piano sociale ed è una negazione e un'offesa del giusto. Dunque, a nome di tutti i cittadini normali e onesti di questo Paese, vi chiedo e vi supplico: abolite i vitalizi, abolite questa vergogna o almeno riducete questa infamia, prima che questa infamia definitivamente vi travolga.

ho veramente difficoltà a separare le bugie dalle sciocchezze in quello che ho testé

ci sono dai sette ai nove milioni di italiani che prendono, come ex statali, una pensione retributiva e non contributiva. Ogni singolo italiano, percepisce circa il 60 per cento in più del monte pensione rispetto ai contributi che ha versato. Se questa fosse una Nazione nella quale nelle Aule del Parlamento non fossero arrivati dei Pulcinella, che parlano senza avere neanche la nozione dell'aritmetica, dovremmo dire che l'istituto delle pensioni figurative, che è uno scempio dello statalismo, ci costa dai 70 agli 80 miliardi di euro all'anno in più. Ora, fare delle questioni sulla vicenda dei vitalizi dei parlamentari per 80 milioni rispetto ad 83 miliardi mi sembra una sciocchezza che solo qualcuno sprovveduto e in perfetta malafede può proferire ai fini propagandistici in questa Aula, nel silenzio annoiato, e purtroppo compiacente

perché uno Stato bolso, ridondante, inefficiente, pauperistico, assistenziale e clientelare da cinquant'anni a questa parte ha utilizzato la leva della spesa a debito crescente. E non lo ha fatto per i propri parlamentari,

dello sperpero e del disastro economico italiano possa essere addebitato a qualche migliaia di parlamentari che godono del vitalizio. Vorrei anche ricordare che i costituenti di allora previdero questa forma di previdenza (che è contributiva, nel nostro caso, e non retributiva, da qualche anno) per dare la possibilità a chi non era di censo elevato, a chi non eserceva una professione liberale, ma che viveva o di un mestiere o aveva un posto di lavoro, di continuare a vivere decorosamente avendo ricoperto l'alta carica di parlamentare della Repubblica. Mi pare che fu il Partito Comunista, attraverso i suoi membri, a dare questa opportunità. Ora, che qualche scalcinato ci venga a dire qua dentro che questa

Vai via! Fammi parlare, deficiente! Fammi parlare!

Dico questo per consegnare al pubblico ludibrio questi rivoluzionari alle vongole, che raccontano frottole e che non distinguono i milioni dai miliardi. Questi piccoli fascisti che non fanno paura a nessuno. *(Proteste

liberale di questo Stato, non rispettando le regole. Quindi lui contraddice totalmente quello che dice di essere e la sua ideologia.

ossia l'equiparazione dei vitalizi del sistema precedente con il sistema contributivo che, come sappiamo, è stato modificato dal Governo nella scorsa legislatura.

Dobbiamo partire da noi perché noi questo facciamo: proviamo a dare l'esempio. Ci tagliamo gli stipendi per dare l'esempio. Io sono salernitano, campano, come sapete, e da noi si dice che il pesce puzza dalla testa. Allora vogliamo ridare un poco di vita e un po' di sano odore a questo pesce? Iniziamo a fare noi qualcosa. qualcosa. Noi abbiamo dei casi, da salernitano purtroppo lo so, di ex deputati e Ministri di questa Repubblica che prendono 9.000 euro al mese di vitalizio da quando avevano quarantotto anni. L'esempio è Pecoraro Scanio tanto per dire nome e cognome. Non penso che sia una cosa bella per i cittadini vedere che avvengono queste cose. E allora perché i cittadini, i pubblici dipendenti, e oggi anche i parlamentari hanno il sistema contributivo e lor signori no? Che cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo di dare l'esempio e lo stiamo chiedendo ai più alti rappresentanti di questo popolo.

E fino a quando ci siamo noi, in un certo senso il dramma e la disperazione della gente trovano la possibilità di essere rappresentati dal Movimento 5 Stelle. Ma se non ci fosse il Movimento cosa accadrebbe?

e ciò non avviene per il Senato, nonostante nella discussione del bilancio dell'anno scorso fu approvato un ordine del giorno, il G29 (testo 2) che prevedeva proprio la pubblicazione dei compensi e dei consulenti del Senato. Questo non è avvenuto quindi con questo ordine del giorno noi chiediamo al Collegio dei Questori e al Consiglio di Presidenza di applicare quando previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

ed ha prodotto tante altre offese, io vorrei rispondere in maniera un po' più signorile dicendo che è un totale ipocrita perché lui insieme a tanti altri che si riempiono la bocca dicendo che occorre diminuire i costi della politica, all'atto pratico sono quelli che hanno contribuito a violentare la Costituzione con il falso obiettivo di ridurre i costi della politica. A tale proposito mi rivolgo al Partito Democratico per dire che questa è la gentaglia con cui state violentando la Costituzione. Ebbene, per quanto riguarda i vitalizi, visto che il collega D'Anna ha parlato anche, offendendo il collega, di Pulcinella senza cognizione dell'aritmetica, io vorrei far presente che che il capitolo riferito al trattamento dei senatori cessati dal mandato, prevede una spesa di 83 milioni di euro per l'anno 2016. Questo era lo stesso importo previsto per l'anno 2015

sono all'oscuro dei cittadini, perché non vengono quasi mai trasmesse in *streaming*. Con questo ordine del giorno chiediamo al Collegio dei senatori Questori e al Consiglio di Presidenza

di una strumentazione idonea a trasmettere via *streaming* tutte le riunioni e anche a potenziare la *web* TV del Senato. Per quanto riguarda l'ultimo ordine del giorno G41 c'è da dire che purtroppo la prassi consolidata in questo Senato ha molto più valore del Regolamento e, per quanto riguarda il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo del Senato, i senatori non hanno possibilità di incidere in alcun modo con gli emendamenti.

Quindi, chiediamo che venga dedicata una sezione specifica del sito *web* del Senato all'*iter* di attuazione degli ordini del giorno, affinché i cittadini possano sapere all'esterno

perché i lavoratori non ne avevano diritto. Avete detto: ci sono tante persone che prendono tanto, ma non ne avevano diritto, perché soltanto negli ultimi anni hanno accumulato tanti soldi e la pensione era calcolata soltanto per gli ultimi anni di lavoro. Questo era il sistema pensionistico basato sul calcolo retributivo. Lo avete attaccato.

e appunto mi domandavo questo: se queste persone stanno dicendo questo, forse io non ho ben capito allora come funzionano la solidarietà il sistema sociale di uno Stato. Forse quando comincerò a studiare meglio, quando sarò più adulto, allora capirò. Gli anni sono passati e credo di essere diventato adulto; ebbene, stavate prendendo in giro ancora una volta gli italiani. Avete distrutto il sistema sociale e l'avete sostituito con un'altra cosa. Avete diffuso il terrore: non avrete più la possibilità di prendere la pensione. Dobbiamo cambiare. Quindi che cosa avete fatto? Avete sostituito il sistema sociale della nostra Carta costituzionale, che in realtà - lo ricordo a me stesso

propria vecchiaia. Ci doveva pensare lo Stato. E invece no, lo avete stravolto, perché poi non c'era neanche nessuno a contrastarvi; il Movimento 5 Stelle non esisteva, eravamo ancora giovani; ma oggi siamo cresciuti e siamo qui, vi stiamo contrastando e chiediamo ai cittadini di aiutarci a contrastare il vostro sistema. Cosa ha creato il vostro sistema? La concezione che quello che era stato dato ai nostri padri, cioè il sistema contributivo pensionistico, non funzionava, per cui bisognava creare un nuovo pilastro. Così lo avete chiamato: il pilastro, il secondo pilastro previdenziale, un nuovo sistema previdenziale che doveva integrare, fare da complemento al sistema previdenziale esistente. A chi lo avete affidato? Giustamente qualcuno potrebbe dire: ovviamente sempre allo Stato. No, lo avete affidato completamente ad un sistema privato; quindi, avete tolto allo Stato per dare a qualcun altro. Però, i vitalizi no, i vitalizi parlamentari ve

Grazie comandante! Vorrei soltanto una esemplificazione su quelle che sono le regole dello svolgimento dei lavori in quest'Assemblea perché poco fa, da quello che ho capito - lo chiedo appunto a lei, che presiede - lei lei ha richiamato all'ordine il senatore Martelli, perché parlava mentre parlava un altro collega, ma il senatore D'Anna, che ha lanciato un *dossier* contro un capannello di persone, non è stato richiamato.

almeno - questo sì che è possibile - chiediamo un ulteriore contributo, ovvero una sorta di equiparazione a quello che è lo stato attuale.

una. L'ordine del giorno G27, che riteniamo molto importante, riguarda invece il fatto che molte volte quando si inizia

grazie a tutti

da soddisfare. Chiediamo quindi che almeno il 50 per cento del *budget* che ogni singolo senatore ha in dotazione rimanga al vecchio Gruppo.

io sarò molto breve, perché devo solo illustrare un ordine del giorno con il quale chiediamo l'impegno alla rinuncia da parte dei parlamentari dell'assegno di fine mandato. Ricordiamo che questo equivale all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo. Noi abbiamo assistito a questa *pièce* teatrale in cui sostanzialmente si diceva che non tutto ricade sui costi della politica, che questa è pura demagogia da quattro soldi. Del resto, lo abbiamo ascoltato da colui che ha definito i nostri 8,5 milioni di elettori (ora anche aumentati) dei pezzenti, quindi chiederei addirittura, a fronte di queste dichiarazioni, che gli venisse completamente tolta qualsiasi tipo di indennità e rimborso, dal momento che per alcune persone questi sono soltanto degli spiccioli. Pertanto, a nome di quei 4,5 milioni di nuovi poveri, di persone che non riescono a fare la spesa,

con questo ordine del giorno chiediamo di mettere i piedi per terra ai senatori e ai parlamentari in genere. Cosa significa mettere i piedi per terra? Significa mettersi nelle condizioni di un cittadino qualsiasi, che sa quanto costa l'utilizzo di un telefono, un litro di latte o un chilo di pane e che, magari con un salario di 1.200 euro al mese, deve mettere insieme la cena con il pranzo e far quadrare i conti, per sé e per la famiglia. dal 2011 i senatori ricevono un rimborso forfetario riferito alle spese generali di 19.800 euro all'anno, per spese telefoniche e spese di viaggio accessorie. Come Gruppo politico abbiamo deciso dal primo giorno di stare con i piedi per terra. In questo momento, in qualità di senatori, ogni mese vediamo accreditarci sui nostri conti personali un bonifico suddiviso in più voci. La cifra «rimborso forfetario» è una cifra considerevole, come dicevo, di 1.650 euro ogni trenta giorni.

se non sia il caso di ridurre la cifra del 50 per cento, per evitare di pesare sulle casse dello Stato, cioè sulle spalle dei nostri cittadini italiani, che sono già grazie a tutti

lo abbiamo devoluto a un fondo di garanzia che aiuta le persone che lavorano nelle piccole e medie imprese. Ogni microcredito erogato produce 2,5 posti di lavoro nuovi, in più, e questo per tutti i cittadini, non solo per quelli di un partito o di una parte politica, tutti i cittadini: è una cosa equa e per tutti quanti. Inoltre, ciò che non spendiamo della cifra destinata alle spese generali - in questo caso i 1.650 euro - lo rendicontiamo attraverso spese certificate. Vi ricordate quanto ci avete preso in giro per i nostri scontrini? Ebbene, gli scontrini servono a questo: a ridare indietro parte

che ci hanno mandato in Parlamento a fare una vera e propria rivoluzione del pensiero e dell'etica, chiediamo a quest'Assemblea di prendere l'impegno di ridurre anche i rimborsi forfetari del 50 Se posso permettermi, signor Presidente, aggiungerei anche che per mettere in campo certe scelte non serve approvare delle leggi, visto che il Movimento 5 Stelle in tre anni ha restituito, tra rimborsi elettorali mai riscossi e resi dei nostri stipendi, oltre 58 milioni di euro, per tutti tutti i nostri cittadini. Lo stesso hanno fatto i nostri consiglieri regionali, i nostri parlamentari europei e i nostri consiglieri comunali. Quindi, potete, anche voi, da domani adottare le nostre regole e dare la prova tangibile di aver capito che questo Paese è bisognoso di prove concrete, al di là degli annunci, dei *tweet* e della

soprattutto voi della maggioranza oggi provate a tirare su la testa. Vi invitiamo a votare secondo vostra coscienza. Qualunque sarà la vostra scelta, anche se oggi le truppe dei giornalisti sembra si siano dati alla macchia, sappiate che verrà puntualmente resa nota ai concittadini; tutti i cittadini, anche quelli che vi hanno votato e che si aspettano da voi un guizzo di coerenza tra ciò che raccontate nelle televisioni e quello che fate in queste Aule.

Signor Presidente, per continuare questa illustrazione, che non dubitiamo sarà commentata qui o altrove come un elenco di solite proposte demagogiche e populiste del Movimento 5 Stelle - lo dico in maniera provocatoria

proposte demagogiche o populiste oppure se, al contrario, al di là di queste definizioni dispregiative, non siano misure ragionevoli che sarebbero apprezzate dai nostri connazionali. L'ordine del giorno G7 prevede che la voce del la voce del rimborso spese per l'esercizio del mandato - che, come sappiamo, viene corrisposto mensilmente a noi senatori per l'importo totale di 4.180 euro, diviso in 2.090

documentata e, possibilmente, pubblicata sulla pagina personale del sito *web* del Senato in relazione al senatore di riferimento. Questa misura farebbe sì che al termine «rimborso» si conferisca un significato concreto: il rimborso è quello che mi viene restituito una volta che do la prova di aver anticipato delle somme (questa definizione ricorda la trappola semantica dei rimborsi elettorali dei partiti, ma questo è un altro ragionamento). Noi proponiamo allora

che per le attività politiche anche sui territori o per fini sociali e culturali, come viene indicato nel nostro Regolamento, siano necessari dei fondi. Non diciamo che tutto debba essere fatto *gratis*, ma questa misura di ragionevolezza e trasparenza sarebbe certamente apprezzata da chi poi chiameremo a votarci alle prossime elezioni. L'ordine del giorno G18 si occupa di un altro tema.

partorito dalla montagna in quel grande dibattito relativo al fatto se fosse giusto o meno che senatori o ex senatori, già attinti da sentenze penali di condanna, fossero meritevoli di percepire il vitalizio. Noi sappiamo che il Consiglio di Presidenza del Senato il 7 maggio 2015 ha partorito questo topolino che prevede, come ricordiamo, non già l'abrogazione per chi viene attinto da sentenze definitive di condanna,

queste somme. Quindi, l'effetto educativo, se così vogliamo intenderlo, o punitivo del privare il rappresentante del popolo che viene meno agli obblighi minimi

accessibile ai cittadini i resoconti integrali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Questori; rendiamoli pubblici diamo un serio esempio di trasparenza e di onestà, anche sotto questo aspetto. Creiamo un *database* delle delibere del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Questori, disponibile alla libera consultazione sul sito *web* del Senato della Repubblica. Dimostriamo in questo che vogliamo applicare la Costituzione e non stravolgerla per fini altri. E veniamo ai fini altri. Noi in realtà abbiamo nel bilancio del Senato delle spese che vanno ben al di là di quelle che vengono vendute come risparmio, qualora si trasformi il Senato in "Camera delle Regioni II". in "Camera delle Regioni II". L'ordine del giorno G8 vuole impegnare il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori ad eliminare dalle voci di spesa ammissibili ai fini del rimborso delle spese per l'esercizio di mandato (che, come sappiamo tutti, riguardano la gestione di un ufficio, l'affitto di locali, le utenze, l'acquisto o la locazione di beni strumentali) quelle destinate ai contributi che i parlamentari dei partiti (non certamente quelli del Movimento 5 Stelle) versano al proprio partito di appartenenza, configurandosi così di fatto una forma occulta di finanziamento pubblico al partito. Il Movimento 5 Stelle, nel rispetto della cittadinanza, che si è già espressa con *referendum*, si è sempre schierato contro contro il finanziamento pubblico dei partiti. La nostra, colleghi, è stata una scelta vincente, ci ha permesso di fare vera politica tra i cittadini, con i cittadini e per i cittadini ed ha anche dimostrato che tale politica, nelle ultime elezioni amministrative, è vincente. Vi Vi prego, non insistete a fare come avete già fatto, affrettandovi ad approvare in tutta fretta la Boccadutri, con la quale vi siete spartiti 45,2 milioni di euro.

la percezione che i parlamentari percepiscano emolumenti non adeguati, chiaramente verso l'alto. Ci sono alcuni parlamentari che ricoprono delle cariche all'interno delle Commissioni, ad esempio le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario. Con questo ordine del giorno chiediamo che siano soppresse le indennità riservate a chi ricopre delle cariche all'interno delle Commissioni, perché crediamo che, con uno sforzo si potrebbe iniziare a dare ai cittadini l'idea che i parlamentari si stiano attivando per ingenerare

ci si dovrebbe sempre chiedere se alla fine questi aiuti non si possano casomai conformare in compiacenze in cambio di gradimento elettorale. G36 invece parte da una considerazione. Attualmente, l'Amministrazione del Senato offre a studenti universitari e postuniversitari la facoltà di fare dei periodi di *stage* formativi completamente gratuiti, stipulati in base a delle convenzioni apposite, che garantiscono la copertura assicurativa ma non garantiscono che a questi tirocinanti sia corrisposta una indennità. C'è una legge del 2012, che ha apportato delle modifiche sostanziali all'istituto dei tirocini formativi attraverso l'introduzione di linee guida nazionali. Queste linee guida nazionali, pubblicate nel gennaio 2013, hanno l'obiettivo di facilitare gli adempimenti per i soggetti promotori e si muovono nel contesto di un documento prodotto dalla Commissione europea nel 2012 dal titolo, appunto, «Un quadro per la qualità tra gli *standard* minimi previsti da queste linee guida c'è anche il riconoscimento di una indennità minima per le attività svolte dai tirocinanti. Con questo ordine del giorno noi chiediamo una cosa semplicissima per

programmi di attività di tirocinio formativo e di orientamento, destinati ai neolaureati più meritevoli, nel rispetto di queste linee guida nazionali e fatto salvo il riconoscimento di una congrua indennità per questi tirocinanti. Arrivo ad illustrare l'ordine del giorno

spesso si è fatto riferimento a precedenti parlamentari. Questi precedenti sono raccolti in un archivio,

questi precedenti parlamentari non dovrebbero essere relegati nel perimetro di un *dossier* coperto da una qualche forma di segretezza, ma dovrebbero resi pubblici o quanto meno disponibili, non solo ai cittadini ma soprattutto anche alle forze parlamentari che si trovano a dibattere i provvedimenti in quest'Aula. Tra l'altro, una dottrina giuridica ha manifestato in tempi recenti una tendenza prevalente a riconsiderare questo problema, dicendo appunto che la segretezza non è opportuna e confligge con la necessità di rendere tracciabile e trasparente l'attività di questa istituzione. Quindi, noi chiediamo, a beneficio della comunità parlamentare e anche per mettere tutte le forze politiche sullo stesso piano (anche quelle giovani) e per ottemperare alle osservazioni di una dottrina giuridica recente, di provvedere alla pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Senato o, quantomeno, sul portale Internet dei senatori,

è relativo alla carica di Segretario Generale del Senato della Repubblica. Abbiamo presentato questo ordine del giorno perché nel panorama istituzionale italiano non esistono altre cariche, oltre a questa, che siano a tempo indeterminato. La Costituzione, infatti, prevede che il mandato del Presidente della Repubblica sia di sette anni e quello del giudice costituzionale di nove anni. Invece, la carica di Segretario Generale è attualmente l'unica posizione pubblica apicale sostanzialmente vitalizia. Essa infatti può essere interrotta soltanto per dimissioni spontanee, per collocamento in quiescenza o per una revoca approvata dal Consiglio di Presidenza. Per questo chiediamo che venga introdotta una modifica che preveda un limite quinquennale del mandato per il Segretario Generale, stabilendo altresì che il conferimento dello stesso non sia reiterabile. Passo ad illustrare l'ordine del giorno G34, che tratta un argomento affine, perché stiamo parlando della temporaneità degli incarichi all'interno della struttura del Senato; anche in questo caso stiamo parlando di posizioni reiterate nel tempo che non hanno un corrispettivo in altre situazioni. Infatti, i Servizi del Senato della Repubblica, soprattutto in tempi recenti, sono stati connotati da un sostanziale immobilismo, che ha visto permanere gli stessi soggetti a capo del medesimo Servizio per un lasso di tempo troppo lungo ed incompatibile con le premesse che ho appena fatto. Per questo motivo l'ordine del giorno anche in questo caso chiede l'introduzione di un limite temporale per tali funzioni, ad esempio per i consiglieri capo Servizio,

è relativo a una questione molto pratica, ossia il fatto che attualmente i senatori

è un formato che non consente l'immediato uso ed inserimento nei calendari

attualmente è già disponibile in formato elettronico, venga messo a disposizione in un formato aperto ed accessibile, quindi che possa dialogare con i normali *smartphone* o *tablet*, in maniera tale da poter inserire immediatamente in calendario ed averlo subito disponibile per tutti. Questa è semplicemente una regola di buonsenso che eviterebbe a tanti di noi di perdere tempo in operazioni già compiute da altri.

un ulteriore capitolo per contributi a fondazioni culturali ad altri soggetti e a terzi (qui non si capisce a chi si riferisca) con ulteriori 195.000 euro.

con l'ordine del giorno G26 si impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a ridurre il contributo previsto in favore dei Gruppi parlamentari nella misura del 20 per cento rispetto alle attuali previsioni. È inutile imporre ai cittadini tanti sacrifici quando invece la politica, che dovrebbe dare il buon esempio, si esenta dal farli. La sobrietà è diventata una merce rara e preziosa. Facciamo in modo che diventai invece la nostra vera caratteristica.

G9 parla di missioni. Abbiamo parlato tanto dei costi della politica e di queste Aule e sicuramente le missioni fanno parte di questo

Quindi nessuno dice che le missioni debbano essere cancellate, anzi, spesso sono fondamentali per comprendere la materia del dibattere. Quello che invece vorremmo porre all'attenzione è il costo della missione in sé. Anche in questo caso, nessuno dice che i senatori devono andare in bettole o in posti non consoni consoni però c'è una via di mezzo, ovviamente. Quindi il fatto di chiedere un tetto e una rendicontazione puntuale delle spese mi sembra il minimo sindacale anche perché,

la differenza è come mangia normalmente e come mangia in missione. Direi che un pasto normale, anche se poi spesso e volentieri in missione non si mangiano pasti normali (e questo chi va in missione davvero lo sa), a maggior ragione dovrebbe essere contemplato. Un tramezzino in autogrill o da qualche altra ha un costo diverso e in tal caso non fa nessun danno il fatto che la gente sappia quanto ha speso un parlamentare in missione. Quindi non vedo per quale motivo non debba essere accolta la richiesta di trasparenza sul sito istituzionale delle spese di missione di ciascuno.

e fare solo il piè di lista potrebbe essere molto peggiorativo.

Ciò vuol dire che a oggi sul sito del Senato non è possibile consultare pubblicamente l'albo dei fornitori. Allora, in nome della trasparenza, con l'ordine del giorno G43 chiediamo

Si potrebbe pensare a una cosa del genere. E poi c'è da dire che fa differenza se si vive a Roma, a Trento o in Sicilia, perché le spese sono diverse.

non bisogna essere demagogici e nello stesso tempo ipocriti, perché a quel punto i cittadini si tengono buoni prendendoli in

C'è una ridondanza, una sovrabbondanza incredibile, e non basta. Addirittura adesso 3.000 comitati del sì e 3.000 comitati del no sono finanziati.

un tema spinoso e difficile, che si inserisce - vorrei ricordarlo innanzitutto a me stessa e poi a tutti - in un contesto ben più ampio che ci parla del Paese che eravamo e che non siamo più.

grandi aggregazioni sociali ed economiche; aveva lavoratori e lavoratrici che, attraverso il lavoro, giungevano al traguardo pensionistico con quel modello di calcolo. Noi sappiamo che

ed è ciò che continuiamo a fare oggi, quando tentiamo di tagliare spesa pubblica improduttiva per salvaguardare una spesa pubblica non comprimibile.

Ci manca solo che noi continuiamo, sulla base di un rigore contabile che abbiamo visto dove ci ha portato, a rimettere in discussione oggi un tema che, nell'attuale fase, produrrebbe ai nostri cittadini una perdita drammatica di potere d'acquisto e di capacità. C'entra qualcosa questo con i vitalizi? Sono cose diverse, ma parlano dello stesso Paese. Vorrei ricordare la spesa che il nostro bilancio dello Stato sopporta per pagare oggi le pensioni a coloro

sì. Non sono per rimettere in discussione quel Paese che era e che non c'è più. So, però, che oggi chi governa deve fare i conti con questo Paese, con l'attuale mercato del lavoro e soprattutto con questa economia. E oggi noi rispondiamo nel nostro tempo delle cose che facciamo. Penso che un contributo di solidarietà da quelle persone si possa ricevere, magari per sostenere alcune iniziative, alcuni interventi specifici. Vengo quindi all'illustrazione di un modesto ordine del giorno che ho inteso presentare - e concludo rapidamente, signor

questo Senato è stato capace di risparmiare 152 milioni di euro. Propongo allora, pur sapendo che un ordine del giorno ha il valore che ha e che non è certo impegnativo per alcun *iter* legislativo - è un impegno che propongo al Senato - di destinare questi risparmi a una delle tante diverse emergenze.

affinché almeno noi possiamo portare un nostro contributo alla soluzione di questo problema. Per tornare, invece, al tema di molti altri ordini del giorno, rispetto, soprattutto, ai collaboratori parlamentari, ripropongo un ordine del giorno che già fu accolto l'anno scorso con l'intenzione di darne seguito. Penso che, quando analizziamo i bilanci di qualsiasi organizzazione, così come di qualsiasi istituzione, non ci dobbiamo dimenticare che parliamo di persone di persone che lavorano e della dignità del loro lavoro. Evidenzio, perciò, l'ordine del giorno che riguarda lo *status* giuridico dei collaboratori parlamentari.

da ogni altra implicazione di ordine economico, venga riconosciuto uno *status* giuridico e lavorativo.

Le cifre appena esposte - *in primis* il minore peso finanziario del Senato sul bilancio dello Stato pari a 152 milioni di euro da inizio legislatura ad oggi - ci dimostrano che la direzione intrapresa verso un contenimento delle spese ha prodotto dei risultati significativi. In qualità di ex Questore della Camera dei deputati riconosco la bontà delle azioni intraprese negli ultimi anni dal Collegio dei Questori e da tutti i Servizi dell'Amministrazione.

Si spende meno, ma soprattutto si spende meglio. È il concetto di qualità della spesa ben espresso dal questore De Poli.

Sul fronte del rendiconto 2015, la spesa del Senato scende per la prima volta sotto quota 500 milioni e si attesta sui 495 milioni di euro. non solo: i dati esposti mettono bene in evidenza gli sforzi compiuti per il contenimento delle spese. Il peso finanziario del Senato sulla finanza pubblica si alleggerisce di 152 milioni da inizio legislatura: questo è il dato numerico più importante, che bene sintetizza i risultati delle azioni avviate dal Collegio dei Questori e da tutta l'Amministrazione in un'ottica di razionalizzazione delle risorse. Mi preme ricordare che, oltre alla minore dotazione (risorse chieste allo Stato) pari a 21,6 milioni di euro all'anno (86,4 milioni di euro in quattro anni), si registrano ulteriori risparmi pari a 65,5 milioni di euro. Sono ulteriori risorse che il Senato risparmia e restituisce alle casse dell'erario. Tra l'altro, in questo mio breve intervento, mi preme sottolineare come per gli impegni contenuti nell'ordine del giorno G1, approvato lo scorso anno in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, il processo sia stato avviato per quello che attiene all'armonizzazione delle discipline che riguardano il personale e i parlamentari (*status* unico dei parlamentari, ruolo unico e statuto unico dei dipendenti) e l'integrazione dei servizi. Ricordo i passi in avanti compiuti nel processo che porterà al modello organizzativo del Polo parlamentare con lo scopo di realizzare sinergie e risparmi, mirando tra l'altro anche a migliorare la qualità dei servizi offerti. Nell'ambito del processo di integrazione funzionale tra Camera e Senato, gli organi di direzione politica delle due Camere hanno premuto sull'acceleratore formulando indirizzi comuni volti a procedere alla definizione di forme di collaborazione, unificazione e integrazione tra le attività delle due Amministrazioni. E ora bisogna portare a compimento questo processo con l'obiettivo di conseguire maggiori risparmi. Per ciò che riguarda le gare, i primi passi importanti in termini di integrazione dei servizi di settori omogenei dei due rami del Parlamento sono stati compiuti. Basti pensare alla gara di prestampa condotta insieme dalle Amministrazioni di Camera e Senato. Ora, però, bisogna spingersi più in avanti, andando verso la centrale unica di committenza. Concordo con il senatore De Poli sulle valutazioni di integrazione con l'altro ramo del Parlamento. La *mission* finale - che non dobbiamo perdere mai di vista - è di modernizzare le istituzioni del Paese. Vanno in questa direzione i passi compiuti finora. Si tratta di un processo che è partito e che riguarderà più campi delle due Amministrazioni e tutto ciò porterà a sinergie e, quindi, a risparmi di spesa significativi. In questo senso, mi preme, infine, mettere in evidenza come sia importante che il processo di unificazione e integrazione venga accompagnato da un percorso di armonizzazione delle regole di contabilità dei due bilanci e dalla redazione di un bilancio integrato, volto a mettere in evidenza i risparmi derivanti proprio dalla riorganizzazione delle strutture e dalla razionalizzazione che ne conseguirà. Vale la pena, infine, ricordare come in un contesto internazionale il Parlamento italiano spicchi per la trasparenza che, non sempre, trova corrispondenza nei Parlamenti di altri Paesi. l'istituzione di Palazzo Madama, ancora una volta, spicca positivamente nel panorama istituzionale per un fatto di trasparenza, oltre che per il *trend* decrescente delle spese considerando che, mentre in generale le spese delle amministrazioni dello Stato

Signor Presidente, vorrei ringraziare l'Ufficio di Presidenza e i senatori Questori per il bilancio che ci hanno presentato. Hanno lavorato con costanza, capacità e serietà, serietà, cercando di contrarre le spese al massimo. Naturalmente in un'organizzazione si guarda se le spese sono state giustificate dalla produttività,

se avessimo razionalizzato meglio i nostri lavori e avessimo sprecato meno tempo, probabilmente avremmo speso meno in luce ed energia, perché avremmo lavorato più proficuamente

razionalizzazione. Ho chiesto, però, la parola a nome di Forza Italia - spero di interpretare anche i sentimenti di tutti i senatori - per fare un ringraziamento veramente sentito nei confronti delle 669 persone che lavorano per noi. noi. Vorrei sottolineare un aspetto che mi sembra importante. Fra pochi mesi - non sappiamo ancora la data, ma si tratta di qualche mese - il Paese si pronuncerà, tramite il *referendum*, sulla riforma costituzionale

Credo, pertanto, che sia giusto ringraziare queste 669 persone che, pur in situazioni psicologiche difficili, hanno cercato di aiutarci nel nostro lavoro. E se abbiamo fatto degli errori, non è certo dovuto a loro carenze.

come sapete, i documenti contabili al nostro esame sono fondamentali per il funzionamento del Senato della Repubblica e - come ha detto il relatore, senatore Questore De Poli, che mi ha preceduto - evidenziano i risultati positivi che abbiamo conseguito negli ultimi e quelli che saranno conseguiti anche nei prossimi sul fronte del risparmio delle spese. Da essi si evince che anche quest'anno il Senato mantiene fermo l'impegno, ormai intrapreso da un po' di tempo, volto a contribuire positivamente alla riduzione della spesa pubblica.

quindi, un progressivo processo di riorganizzazione sia del personale che dei servizi; un processo di riorganizzazione che ha consentito, nel contempo, di garantire a questo ramo del Parlamento lo svolgimento delle funzioni democratiche con precisione e approfondimento, grazie anche alla dedizione che il personale ha messo nel suo lavoro.

si è conseguito un risparmio di spesa per il funzionamento del Senato pari a circa 152 milioni di euro, di cui 86 circa per minore dotazione e 66 per effetto di somme restituite. Nel solo 2015 i risparmi conseguiti sono stati pari a 5,8 milioni di euro. Il tetto alla retribuzione dei dipendenti porterà poi a regime ulteriori risparmi per circa 36 milioni di euro. Altri 31 milioni di euro di risparmi derivano dal contenimento - anche quello c'è stato - delle indennità parlamentari e delle competenze accessorie. Venendo al merito dei documenti, mi limiterò a evidenziare soltanto alcuni dati che mi sono sembrati più significativi.

E se si allarga l'orizzonte a partire dall'inizio della legislatura, la spesa effettiva del Senato si è ridotta del 4,83 nell'anno 2015 si conferma da parte del Senato la restituzione allo Stato, sulla base di un decreto-legge che abbiamo convertito in legge nel 2014, dell'importo complessivo dei risparmi realizzati nel corso degli esercizi finanziari; insomma, sono state liberate risorse che possono essere utilizzate

È stato poi fatto riferimento al contributo di solidarietà, anche questo a carico dei trattamenti pensionistici degli ex senatori e degli ex dipendenti, pari a circa 7 milioni di euro per il 2015, che sarà restituito alle casse dello Stato. poi sottolineare che, negli ultimi anni, sono costantemente diminuite le voci relative ai rimborsi di natura indennitaria per i senatori in carica, nonché le somme erogate per i senatori cessati dal mandato. Drastiche riduzioni si registrano, nel 2015, sul versante dei costi per il trattamento del personale dipendente, che in termini assoluti passa da 119,3 milioni di euro nel 2014 a 102,4 milioni

Un consistente contributo alla riduzione della spesa di funzionamento deriva dalla voce relativa alla spesa per il personale dipendente, che è prevista diminuire di circa 2,2 milioni di euro, Le spese in conto capitale sono previste in leggero aumento rispetto a quanto preventivato nel 2015. Per quanto riguarda le entrate, l'unico dato rilevante riguarda il differenziale relativo al Fondo iniziale di cassa, che scende da 13,155 milioni di euro del 2015 a 12,355 milioni di euro nel corrente anno. Nel complesso, quindi,

Preso atto dei risultati conseguiti nel corso degli ultimi anni, credo che sia nostro dovere proseguire nello sforzo di razionalizzazione e di efficientamento dell'istituzione Senato. Ritengo che sia questo il giusto contributo che la classe politica deve offrire alla collettività. E deve essere uno sforzo da compiere al netto dell'esito del percorso della riforma costituzionale. In questo auspico due fondamentali passaggi nel prossimo anno: il completamento del percorso relativo al ruolo unico del personale dipendente

al prossimo anno ed è necessario intervenire in questa direzione, per revisionare e migliorare ulteriormente la spesa del Senato.

grazie a tutti

grazie a tutti

togliendo quanto resta, perché è inutile avere un canale per ogni Commissione quando i lavori delle Commissioni in genere non possono essere pubblici. Abbiamo già otto canali per la trasmissione della *web* tv e in questo momento sono addirittura sovrabbondanti rispetto alle possibilità di fare trasmissioni pubbliche dei lavori delle Commissioni.

per la pubblicazione di delibere del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Questori di interesse generale». Non può essere una cosa generalizzata perché ci sono alcuni aspetti, anche delicati, che riguardano gare di appalto che non possono essere anticipate all'esterno prima che il Consiglio di Presidenza, per esempio, abbia accettato quanto proposto dai Questori, ma con questa formula siamo favorevoli. Esprimo parere favorevole

del giorno G45 come raccomandazione, in quanto da parte nostra ci possiamo attivare per poter avere il collegamento con le banche dati del Ministero dell'economia, ma tale Ministero deve renderle disponibili. Ricordo che proprio la settimana scorsa, esaminando il disegno di legge sugli enti locali,

se la senatrice Comaroli accogliesse una piccola modifica che riguarda coloro che sono stati buttati fuori dal Gruppo. Ci sono persone che hanno scelto liberamente e persone che, in modo irregolare, illegittimo e non giustificabile, sono state estromesse dal Gruppo con cui sono legittimamente entrate. Per la verità, questi avrebbero anche diritto a un risarcimento,

Il tema che ha sollevato la collega Comaroli è un tema di grande rilevanza per lo svolgimento della funzione parlamentare, in special modo per la funzione importantissima e delicatissima che svolge la Commissione bilancio.

che, in teoria, dovrebbe consentire a tutti di accedere a quel dato. Vedo che ci sono colleghi che conoscono bene la dinamica di questa problematica e sanno che questo non vuol dire quasi niente. Il punto è che accedere al *data mart* che consente di verificare la copertura e la reale esistenza del fondo grazie a tutti la volontà del Ministero dell'economia e delle finanze che, evidentemente, non è ancora stata registrata positivamente in ordine a questo; dall'altro, il problema è implementare quella struttura

anche impossibile per la Commissione bilancio poterlo avere nel tempo reale che serve per fornire le coperture finanziarie necessarie quando i colleghi presentano emendamenti che la Commissione deve valutare in modo autonomo e indipendente dal Ministero dell'economia

una tendenza alla contrazione delle spese. Passiamo infatti dai bilanci che oltrepassavano i 650 milioni a questi che sono sotto i 500 milioni.

Stiamo soltanto aspettando ad ottobre un verdetto popolare che sancirà se il Senato s'ha da chiudere o non s'ha da chiudere. Cosa succederà se chiuderemo questo Senato? Qualcuno potrebbe dire che risparmieremo

Cosa risparmierebbe un cittadino italiano se dovessimo chiudere il Senato? Prendendo la cifra di 495 milioni, ogni cittadino risparmierebbe 0,67 centesimi ogni mese; lo ripeto, risparmierebbe mezzo caffè ogni mese. Ma non è giusto, non è così, perché abbiamo il bilancio abbastanza dettagliato e vediamo come è ripartito: 102 milioni sono per il personale dipendente. Ancorché noi chiudessimo il Senato, non credo che si possa sopprimere il personale, che verrà dislocato in altri enti, verrà ripartito, quindi queste spese non potranno essere cancellate. per i 10 milioni del personale adibito alle segreterie della Presidenza e via dicendo. Come non possono essere cancellati i 138 milioni per i dipendenti in quiescenza. Non possiamo andare a casa

giusti o sbagliati che fossero, i vitalizi degli ex senatori, che ammontano a quasi 80 milioni. L'unico risparmio che, chiudendo il Senato (ancorché non sarà così perché i nuovi senatori avranno lo stesso dei costi, riceveranno delle indennità

Questo significa che i numeri che ho dato prima non valgono più, perché ogni cittadino italiano si vedrebbe nelle proprie tasche, dato il risparmio, un aumento di ben 13 centesimi a testa. Lo ripeto perché rimanga agli atti: ogni italiano risparmierebbe 13 centesimi al mese. Allora abbiamo capito cosa sono i costi della democrazia.

Non sono invenzioni, ma i dati che emergono analizzando questo bilancio. Se poi dovessimo fare un altro conto parallelo, per cui per ogni immigrato

la cifra del Senato ammonterebbe a nemmeno la metà dei costi per l'accoglienza: i costi della democrazia sono - ripeto - meno della metà dei costi dell'accoglienza. Bene, noi apprezziamo il lavoro fatto dai senatori Questori, apprezziamo il *trend* della revisione della spesa, apprezziamo i risultati concreti che abbiamo visto nell'arco della scorsa legislatura, continuati anche in questa legislatura. Il mio Gruppo dice che non possiamo entrare troppo in questo bilancio, perché non abbiamo un senatore Questore e non abbiamo la possibilità di incidere nelle scelte. Non ci sentiamo più di tanto di criticare queste scelte, pertanto annunciamo una benevola astensione da parte della Lega Nord.

per noi positivi perché si inseriscono all'interno di quella importante scelta che il Consiglio di Presidenza ha effettuato sin dal 2013, cioè quella di razionalizzare le spese e tentare di eliminare gli sprechi in modo da ridurre i costi generali del Senato senza però farne venir meno la funzionalità.

consideriamo questo lavoro abbastanza positivo. Tutti noi oggi abbiamo avuto modo di poterli leggere. Tuttavia credo sia doveroso rispondere anche ad un vecchio insegnamento che impone che i numeri devono cantare politica, quindi dobbiamo aggiungere una lettura politica a questi numeri. Tante cose sono state dette e tante cose sono state scritte sui costi eccessivi del Senato. I populismi di questi tempi, sia quelli di maggioranza che quelli di opposizione, sbandierano continuamente dati a sostegno di tesi contrapposte.

una delle motivazioni che hanno contribuito ad allontanare i cittadini dall'avere fiducia e stima nei propri rappresentati. Oggi non possiamo ignorare che sia in atto un processo di razionalizzazioni e forti cambiamenti che ovviamente incontrano mille difficoltà ma che il Senato sta portando Tutto ancora troppo lento, sicuramente, ma non era per niente scontato riuscire a fare risparmi seri al Senato e per di più con una scelta presa da tutta l'Assemblea legislativa. Credo che noi dovremmo riuscire a spiegare bene tutto questo ai cittadini, dovremmo spiegarlo con chiarezza e trasparenza perché purtroppo negli ultimi tempi ascoltano autorevoli esponenti del Governo, a partire dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per le riforme, che fanno riferimento agli importanti risparmi economici che deriverebbero con l'approvazione della riforma costituzionale che non elimina il Senato ma elimina solo il diritto di scelta e di partecipazione dei cittadini. Dopo aver mandato a casa 3.000 politici ora lo *spot* governativo è dare un calcio ai 315 senatori. A parte il cattivo gusto e il poco dignitoso silenzio dei colleghi della maggioranza, vorrei far notare che il bilancio del Senato è diviso in due macro aree: il 54,88 per cento, cioè 272 milioni, serve per le spese di funzionamento per cento, cioè 223 milioni, per le spese di natura previdenziale. Nelle spese di natura previdenziale sono compresi i costi dei senatori, del personale dei Gruppi, dei dipendenti e gli oneri I costi delle competenze dei senatori, lo ha detto il senatore Divina prima, ammontano a circa 41 milioni, dunque il risparmio del Senato con la riforma potrebbe essere di 41 milioni perché il Senato dei nominati continuerà a funzionare e avrà i suoi costi. Non vorremmo, tuttavia, aggiungo una riflessione, trovare questo risparmio, ovviamente in quota parte al numero di 100, nei bilanci a carico delle Regioni. Non credo infatti che si risparmieranno i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del mandato. I prossimi senatori, pur nominati e anche solo 100, avranno doppio Non credo risparmieremmo i famosi vitalizi dei senatori eletti prima del 2012 perché, come la discussione di oggi ha dimostrato, è un tema delicato, siamo nel campo dei diritti acquisiti ma sarebbe molto interessante e utile trovare una seria soluzione al sistema pensionistico di tutti i parlamentari, trovando le strade per riportare tutto e tutti nel sistema previdenziale ordinario, un tema complesso che richiederebbe attenzione e forse anche un altro presidente dell'INPS con cui confrontarsi. Non credo si risparmieranno i trasferimenti ai Gruppi parlamentari, perché nonostante non si sappia ancora se il prossimo Senato avrà i Gruppi parlamentari, presso i Gruppi lavorano tantissime persone, molte precarie da anni (i famosi precari storici), lavoratori e lavoratrici ascritti alla delibera del 1993. E questo vale anche per i lavoratori e le lavoratrici delle segreterie. E non credo che si vorrà risparmiare il costo del personale dipendente con

grazie a tutti Ma è necessario e doveroso e non più rinviabile trovare a questo tema una soluzione: si chiama giustizia sociale. Da tempo, prima della riforma costituzionale, è in atto un lavoro di unificazione del ruolo dei dipendenti e dei parlamentari di Camera e Senato per la costituzione del ruolo unico. Un lavoro ancora *in fieri*, ma mi permetto di segnalare a noi tutti che dobbiamo avere tutela del personale dipendente e anche di tutti i precari che sono parte integrante da anni del Senato. Infine, vorremmo ringraziare per il loro lavoro, professionalità, dedizione e passione, tutti i dipendenti e le dipendenti del Senato, il Segretario Generale, i Vice Segretari Generali, i dirigenti, i funzionari, gli assistenti parlamentari, gli stenografi, gli archivisti, i bibliotecari, i funzionari addetti alle votazioni, grazie a tutti per l'alto senso dello Stato che ogni giorno consegnano a noi tutti.

ma perché è il sostantivo più appropriato per descrivere un bilancio che dovrebbe rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria del Senato e che, invece, grazie alle scelte di questa maggioranza, è un documento privo di attendibilità. Le ragioni delle nostre accuse sono varie e alcune di esse hanno anche origini lontane. Infatti, come ripetiamo ormai da tre anni, la mistificazione della realtà contabile del Senato è cominciata nel 2013, allorché, al fine di raggiungere i risparmi previsti dall'ordine del giorno G100 del 2011, grazie a un artificio contabile, vennero spostate tra le partite di giro somme che in tutti i bilanci precedenti erano erano sempre state collocate diversamente. Quello spostamento di capitoli di bilancio, in poche parole, fu fatto al solo scopo di far apparire un risparmio di 20.300.000 euro che in realtà non c'era. La truffa del bilancio del Senato è poi proseguita anche nel 2014 continuando a inserire tra le partite di giro i contributi a favore del Fondo di previdenza del personale del Senato e i contributi a favore del Fondo di solidarietà fra i senatori. Se queste voci fossero state lasciate lì dove erano sempre state fino al 2012 avremmo avuto spese maggiori di oltre 20 milioni di euro rispetto a quelle dichiarate.

al trucco di spostare nei fondi di riserva le somme ridotte dai capitoli di spesa in modo da poter affermare, a chiacchiere, di aver fatto dei risparmi mentre, in realtà, c'è stato solo uno spostamento contabile. Quest'anno i fondi di riserva sono aumentati di ben 500.000 euro rispetto all'anno precedente. Entrando nel merito dei singoli capitoli, possiamo notare che il Senato prevede di sperperare sperperare 1.965.000 euro per spese di cerimoniale e rappresentanza, alle quali vanno aggiunti i contributi a misteriose fondazioni e a terzi per 195.000 euro e i contributi per il fantomatico circolo di Palazzo Madama per 50.000 euro. Come se non bastasse, inoltre, anche su questo bilancio grava ancora il costo per il rinnovo annuale del contratto con RAI Way, per la modica cifra di 400.000 euro: soldi letteralmente regalati, o meglio, buttati solo per il disinteresse e la negligenza del Ministero dello sviluppo economico che, nonostante la previsione esplicita dell'articolo 14*-bis* della legge n. 221 del 2012, non ha ancora preso i provvedimenti necessari per consentire la trasmissione dei nostri lavori sulla piattaforma gratuita del digitale terrestre. Un altro esempio di contabilità creativa è è relativo all'avanzo di esercizio, ovvero quell'importo che si forma con l'approvazione del rendiconto, quando vi sono minori spese o maggiori entrate rispetto a quelle preventivate. Tuttavia, la singolarità del Senato è data dal fatto che ogni anno, tra il bilancio di previsione e i dati finali del rendiconto, si formano avanzi di esercizio molto rilevanti, e anche quest'anno assistiamo a un avanzo d'esercizio di ben 44.222.684,79 44.222.684,79 euro. Questa somma viene solo in parte riportata nel bilancio di previsione 2016, e infatti nel fondo iniziale di cassa ritroviamo solo 12.355.146 12.355.146 euro. La scelta di ripartire su più anni gli avanzi d'esercizio è incomprensibile dal punto di vista logico e contabile; sicuramente non aiuta nella chiarezza e nella trasparenza, tant'è vero che ogni anno si deve richiedere appositamente all'Ufficio di ragioneria il prospetto con le quote residue di avanzi d'esercizio di anni precedenti non ancora utilizzate. Vi sono ancora significativi margini per la riduzione della spesa del bilancio e, quindi, della dotazione che il Senato riceve dallo Stato. Ma è ormai abituale prevedere spese superiori. superiori. La verità è che se le previsioni venissero fatte in modo più obiettivo, le risorse che lo Stato versa al Senato potrebbero essere ridotte, ma tanto a noi non c'importa, perché mica noi siamo lo Stato! Noi del Movimento 5 Stelle nello Stato ci crediamo ancora e, quindi, il nostro voto sarà contrario.

il *referendum* ha come obiettivo quello di mettere in atto un risparmio, per lo Stato importante e utile - che tutti vogliamo perseguire - la relazione che abbiamo sentito oggi dai Questori dimostra che questo risparmio il *referendum* non lo otterrà in maniera così importante da essere uno dei motivi per cui è giusto appoggiare il cambiamento costituzionale.

Con i dati che abbiamo preparato vogliamo sottolineare che, se l'obiettivo che si persegue con le riforme costituzionali è quello di ottenere un risparmio, conti alla mano, questo risparmio non lo otterremo.

continuo miglioramento della trasparenza e di questo sicuramente i cittadini saranno contenti. In questo senso, nel manifestare la nostra soddisfazione per l'andamento virtuoso della spesa dell'Amministrazione, dichiaro il voto favorevole del Gruppo FI- PdL XVII, sia sul rendiconto che sul bilancio di previsione,

sia stato un momento apprezzabile di confronto e che quando un'istituzione approva il proprio bilancio non compie semplicemente un atto che serve a rispettare regolamenti e procedure, ma vive un momento politico di alto livello: il dibattito, infatti, ha toccato

però che le motivazioni non abbiano trovato il giusto orgoglio, la giusta rivendicazione da parte di quest'Aula. In sintesi vorrei quindi riproporre quali

ma in questo caso, che la massima istituzione dello Stato, in un momento in cui chiediamo tutti insieme sacrifici al Paese, si sia impegnata costantemente negli ultimi anni su un percorso di riduzione dei costi e abbia mantenuto questi impegni, fatto da rimarcare con grande soddisfazione. In particolare dal 2006 ad oggi il Senato rappresenta, nell'ambito dei costi della pubblica amministrazione, lo 0,06 per cento rispetto allo 0,083 di allora. grazie a tutti dire se l'efficienza e l'efficacia dell'istituzione che rappresentiamo sia stata raggiunta in senso pieno; lo diranno i cittadini. Tuttavia questo primo aspetto simbolico credo sia un merito raggiunto, come lo è - lo ricordava il senatore Tonini - aver tenuto il punto su quello che l'ordine del giorno G100 dettava come un traguardo che allora poteva sembrare ambizioso. Con il lavoro di tutti gli anni, portato avanti dal Consiglio di Presidenza e dal Collegio dei senatori Questori, abbiamo mantenuto questo ritmo di tagli, ma preservando l'efficienza e il funzionamento del Senato. Sicuramente, come hanno già ricordato in molti, questo va in gran parte riconosciuto come merito al personale dipendente, a cui sono stati chiesti i maggiori sacrifici in termini di riduzione del peso all'interno del bilancio del Senato, senza che venisse meno la qualità del servizio. Tutti insieme abbiamo sottolineato come ciò significhi una sola cosa: alta professionalità. Dobbiamo quindi riconoscere loro questo merito e anche quello di accompagnare con grande senso di responsabilità anche la loro rimodulazione contrattuale. Qualche volta è importante dire ai cittadini che stiamo facendo bene, che lo stiamo facendo insieme e lo considero importante anche per le forze di opposizione. Qualche ordine del giorno è stato definito ironicamente demagogico; non credo che lo siano stati tutti, ma sicuramente è demagogico nascondere i successi di cui dobbiamo andare fieri. Per quanto riguarda i tagli - e chiudo - è evidente che abbiamo portato la macchina a un livello di efficienza molto significativo. Così come è evidente a chi vuole perseguire tagli più ragguardevoli, come quelli che sono stati indicati, che solo la riforma costituzionale consentirà di raggiungere questo risultato. Per quanto ci si affanni e ci si sia affannati nel voler ricostruire dati che minimizzano il risultato di quei tagli, è chiaro, già dalla lettura di questo bilancio, come dalla sola voce dei senatori si ottengano risparmi di un ordine di grandezza superiore a quello di cui oggi ci stiamo rallegrando. È chiaro altresì che, andando a regime la riforma, questi risparmi aumenteranno, anno per anno. Infatti tutti i progetti ambiziosi hanno bisogno di anni per andare ad assestamento. Ma soprattutto è chiaro che i risparmi più importanti che doneremo agli italiani non saranno solo quelli del bilancio del Senato, ma saranno quelli delle inefficienze che verranno meno, portando le Regioni e le autonomie a Roma nel momento legislativo e avviando un processo legislativo più rapido,

*(M5S)*. Signor Presidente, sono passati ormai mesi, se non anni, dal giorno in cui si parlò in maniera più precisa della terra dei fuochi. dei fuochi. In quel periodo, siccome c'era attenzione mediatica e, quindi, i telegiornali davano una certa attenzione a chi parlava di quel problema, problema, il presidente del Consiglio, mai votato dai cittadini, Renzi fece un annuncio e venne anche a Napoli (ovviamente fischiato perché il popolo napoletano non si fa prendere per il naso)

c'è di mezzo la vita dei cittadini. La terra dei fuochi brucia ancora; purtroppo sono giorni che nella Provincia di Napoli vengono bruciati roghi. L'ultimo, purtroppo, è stato accesso purtroppo, è stato accesso sul Vesuvio. Probabilmente non si tratta di rifiuti, ma comunque questi balordi ancora stanno a piede libero. Con quei soldi bisognava invece verificare e monitorare il territorio. Noi chiediamo al Ministro nuovamente un tavolo immediato affinché venga nuovamente finanziato un intervento per la terra dei fuochi al fine di debellare questi porci e balordi.

ho solo espresso un'opinione in cui credo proponendo l'ordine del giorno per l'abolizione o, quantomeno, la decurtazione dei vitalizi. Il senatore D'Anna può avere un'opinione diversa e poteva esprimerla senza offendere nessuno.

insieme al vicino di banco, ci ha deliziato con le simulazioni sessuali. Ricordo anche quando, utilizzando una frase di Al Capone, riferendosi proprio a lei ha commentato: «È solo chiacchiere e distintivo», paragonandola a Ponzio Pilato e chiedendo le sue immediate dimissioni per manifesta incapacità. Dopodiché ha iniziato uno sciopero della fame che non ha ancora concluso (però a guardarlo non mi sembra abbia effetti). *(Ilarità).* A parte questi miei ricordi - e invito il senatore D'Anna a continuare ad attaccare la mia persona o il Gruppo perché sarò fiero

queste parole già ci siano. «Manfrina mendace», sì va bene; «Pulcinella», rivolgendosi a tutto il Gruppo; a me personalmente «scalcinato», «sprovveduto», in «malafede» e «deficiente», rivolgendosi al Capogruppo; «rivoluzionari alle vongole» e «piccoli fascisti» a tutti noi; «pagliaccio», rivolgendosi al senatore Cioffi. Oltre a queste parole, che ricordo a memoria, si è permesso addirittura di lanciare prima un foglio e poi, non contento, un fascicolo al senatore Lucidi. Signor